trovo leggermente paradossale - per usare un eufemismo - che la maggioranza si preoccupi (è una preoccupazione legittima) che domani mattina possa riferire il Ministro dell'interno sugli accadimenti delle piazze italiane e non sia più urgente il fatto che, prima del ministro Lamorgese, venga a riferire in questa Assemblea il presidente Conte, che è il responsabile politico di quanto sta avvenendo nelle piazze italiane. A noi fa piacere che il ministro Lamorgese venga a dirci qual è stato l'operato delle Forze di polizia, cui va la nostra totale solidarietà, però prima è è importante che nella casa degli italiani, cioè il Parlamento, venga il primo ministro Conte, che si è preso quattro giorni di tempo per riferire su questioni urgentissime e drammatiche per la vita di centinaia di migliaia

Al tempo stesso, ringrazio il sottosegretario Laura Agea per il tratto di signorilità che ha contraddistinto il suo operato in seno alla 14a Commissione, di cui sono onorata di fare parte.

In particolar modo, ringrazio il collega, senatore Pittella, che ha messo sempre a disposizione la sua esperienza in un rapporto di stretta collaborazione. Signor Presidente, tutto ciò assume una valenza particolare visto che ancora oggi la pandemia ci attanaglia, ci spinge e ci sollecita a rapporti di collaborazione per mettere insieme tutte le nostre energie, le nostre forze,

una nuova finestra"). Comunico che sono pervenute alla Presidenza le seguenti proposte di risoluzione, i cui testi sono in distribuzione:

Signor Presidente, relativamente alle proposte di risoluzione, il Governo esprime parere favorevole alla risoluzione di maggioranza e contrario alle altre risoluzioni. Per prima cosa mi corre l'obbligo di fare alcuni ringraziamenti, in particolare alla 14a Commissione del Senato, che ormai da circa un anno lavora alacremente, con grande convinzione e con l'obiettivo di raggiungere il massimo risultato, alla legge di delegazione europea. Nello specifico, il mio primario ringraziamento va al relatore, senatore Gianni Pittella, che con uno spirito di grande collaborazione ha gestito il lavoro in seno alla 14a Commissione, e a tutti

Implementare, in un momento come questo, la normativa europea in seno all'ordinamento nazionale non è cosa semplice, richiede particolare attenzione. Richiede

27 Stati membri, che molto spesso hanno realtà, situazioni e condizioni diverse. Non è stato sicuramente facile trovarci ad implementare nella legge di delegazione europea 2019 un numero così alto di direttive e regolamenti, ma il massimo sforzo che la Commissione e i senatori hanno fatto ci consente oggi di poter dire di essere estremamente orgogliosi e soddisfatti non solo di poter licenziare un testo

di rendere quella normativa adatta e assolutamente efficace con riferimento all'attuale realtà economica e sociale del nostro Paese. di estrema difficoltà, una crisi pandemica alla quale non eravamo preparati, ma che con coraggio e con convinzione stiamo cercando di affrontare anche con questo strumento, cercando di dare attuazione alla normativa europea e di farlo in maniera che essa non gravi troppo sul nostro tessuto produttivo. Non entrerò nello specifico di tutte le direttive e i regolamenti ai quali si dà delega al Governo per la loro attuazione. Mi preme però ricordare come l'Italia oggi ponga Grazie

che regola l'equilibrio tra vita familiare e vita lavorativa, ci consente di dare supporto e sostegno maggiore a quelle famiglie che vivono l'esperienza lavorativa, ma che hanno bisogno di modellarla

la direttiva sul *copyright*, un tema estremamente complesso, sul quale era necessario porre ordine ed attenzione e sul quale l'Italia sta facendo un passo avanti. Credo che l'Italia sia uno tra i pochi Paesi che darà completa attuazione alla direttiva sul *copyright*, cercando anche di dare sostegno e supporto a tutte quelle categorie che, per un motivo o per un altro, fino ad oggi sono state escluse da questa regolamentazione. C'è poi la direttiva sulle fonti rinnovabili: oggi l'Europa parla di *green deal*, di transizione verde, di raggiungimento di obiettivi di neutralità energetica al 2050. Ebbene, questa direttiva va in quella direzione, quella direzione, consente al nostro Paese di fare un passo in avanti, di cercare veramente, anche alla luce di quelle che poi saranno le risorse del *recovery fund*, di andare verso l'ottica della transizione verde, una transizione che ha bisogno di coraggio, che ha bisogno di coraggio, di decisioni importanti, che avranno un impatto forte. Non dimentichiamo che all'interno di questa direttiva parliamo delle comunità energetiche, di quei cittadini che da oggi avranno la possibilità di produrre, stoccare e vendere l'energia. *(Applausi)*. Questi sono passi in avanti. L'Europa sostiene questi cambiamenti. Le energie rinnovabili sono un cambiamento necessario ed una strada da percorrere con coraggio e senza un minimo tentennamento. Mi soffermo brevemente anche su altri argomenti sui quali oggi si pone l'attenzione: la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Quando abbiamo iniziato a lavorare su questo documento, non immaginavamo quanto sarebbe successo di lì a poco, nessuno si aspettava che il mondo, l'Italia, l'Europa si sarebbero trovati a misurarsi con quello che è probabilmente uno degli eventi più inaspettati e tragici dal secondo Dopoguerra. La pandemia ha posto l'attenzione su quelli che devono essere gli obiettivi, i compiti, i ruoli, gli sforzi e le sfide che da oggi in avanti ci troveremo ad affrontare relativamente a tutti i futuri cambiamenti che accadranno dopo la pandemia. Oggi ci troviamo in un momento che ci pone di fronte all'assoluta necessità di ripensare al contesto europeo, alla luce di quelli che saranno cambiamenti che non potremo fare a meno di considerare tali.

Non sono cambiate le nostre priorità, perché già prima della pandemia e parlando dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ci ponevamo interrogativi importanti, erano quelli delle sfide verso una transizione verde, verso la transizione verso il digitale, sfide che dovevano riguardare l'inclusione sociale, un pilastro sociale non semplicemente negli enunciati, ma nella sua concretezza. fondamentale affrontare qualunque tipo di intervento tenendo presenti e saldi questi principi. Credo fortemente che l'impegno del Governo e il mandato forte che il Senato darà al Governo su questi temi ci permetterà di essere credibili in Europa e di portare avanti con coraggio le nuove sfide, i nuovi obiettivi ci pongono di fronte a un interrogativo fondamentale. Noi oggi ci troviamo a programmare, a pensare e a progettare un Paese che dobbiamo lasciare in eredità ai nostri figli e ai nostri nipoti e dobbiamo avere il coraggio di farlo in maniera tale che sia un'eredità della quale essere non solo orgogliosi, ma anche fieri e che renda il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti all'altezza della loro bellezza. *Green deal*, transizione digitale, economia verde, inclusione sociale sono parole che diventano atti concreti non solo

in questo momento emergenziale; qualcosa che possa diventare un moltiplicatore positivo. Il *recovery fund* è diventato un progetto comune; mai l'Europa aveva parlato di un fondo le cui risorse finanziarie fossero recuperate sui mercati con una garanzia posta da tutti gli Stati membri. Io credo che questo sia un passo in avanti e questo deve renderci ancor più responsabili nell'utilizzo di queste risorse: 750 miliardi sono un punto di partenza, ma possono essere un moltiplicatore positivo laddove l'azione di programmazione e il senso di responsabilità impegnino tutti al loro utilizzo non come se fossero nostre risorse, ma come se fossero risorse da lasciare a qualcuno che verrà dopo di noi di noi e che, come noi, saprà non solo utilizzarle ma moltiplicarle, non semplicemente perché siamo bravi a fare le cose, ma perché abbiamo una capacità di ripensare e progettare il nostro Paese da qui e per i prossimi trent'anni. Ringrazio di nuovo il senatore Pittella, la senatrice Gaudiano e i commissari che hanno lavorato con i loro emendamenti, con il

per la presentazione di eventuali emendamenti ad essa riferiti. Il voto finale sul disegno di legge di delegazione europea, la votazione degli eventuali emendamenti presentati alla proposta di risoluzione n. 1,

Grazie

di tutte le leggi europee sull'ordinamento italiano (e ovviamente sull'ambito economico e sociale italiano) prima di recepirle. Questa risoluzione è stata approvata da quest'Assemblea a dicembre 2018. In coerenza con tale testo, abbiamo presentato l'emendamento che prevede semplicemente di chiedere che, per quanto riguarda la legge di delegazione europea, ad ogni singolo provvedimento sia allegato, da parte del Governo, lo studio di impatto

sul contesto italiano. Sembra quantomeno bizzarro che questa cosa non si voglia fare, perché, al di là della posizione politica di ognuno,

la legge di delegazione europea è ormai una sorta di tabù e quindi qualunque cosa possa non rispondere al modello di totale

relativamente agli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8 il Governo esprime un parere contrario. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G1.100,

la prolusione - proprio del Governo - rispetto a quanto sia importante questo disegno di legge di delegazione europea e di recepimento delle direttive, soprattutto per le generazioni future. Ecco, davanti a dichiarazioni del genere, ci saremmo aspettati piuttosto, da parte del Governo, una presa di coscienza rispetto al fatto che oggi andiamo a

presentati chiedono semplicemente di non andare a pesare ulteriormente - a causa delle suddette direttive - sugli impegni di spesa degli imprenditori e di tutti coloro che si occupano di doverle recepire e far rispettare. Poteva essere l'occasione - oggi più che mai - di dimostrare veramente l'attenzione che questo Governo vorrebbe avere avere nei confronti di chi fa attività e di chi produce. Quindi, c'è assolutamente un grande e grave ossimoro tra quello che il Governo dice e quello che fa.

ad ascoltare il perché e il per come del presidente del consiglio Conte che, invece, va avanti senza ascoltare il Parlamento, salvo ascoltarlo il giorno dopo aver preso posizione. Questa era un'ulteriore occasione per poter dimostrare la buona fede e la buona volontà dell'Esecutivo. Dobbiamo prendere atto che il Governo fa delle affermazioni, ma poi va esattamente nella direzione contraria agli interessi degli italiani.

Presidente, essendo precluso l'emendamento 1.7, mi limiterò alla dichiarazione di voto sull'emendamento 1.8 che, per materia, è assolutamente coerente. Signor Presidente, inorridisco per la votazione che si è appena tenuta. Inorridisco per l'argomento e per l'asprezza che ha dimostrato il Governo rispetto alle motivazioni sottese agli emendamenti 1.6 e 1.7. Non è possibile fregarsene dei costi che caleranno sugli italiani e sulle imprese nel momento in cui si approva una normativa. Non è possibile! In questa sede abbiamo chiesto in maniera esplicita al Governo di tenere conto dei costi, della valutazione rigorosa di impatto, della sostenibilità economica e di prevedere un fondo adeguato a sostenere i costi di adeguamento ricadenti sulle attività produttive. Non è possibile che, in parallelo, in 14a Commissione ci sia un parere di maggioranza che scrive esattamente queste cose, ma se le stesse vengono dette dalla Lega, la proposta viene bollata e respinta. Questo vuol dire non considerare l'interesse degli italiani, ma dividere gli italiani!

i nostri bambini, i nostri adolescenti da quei pericoli, di cui vediamo le conseguenze. Gli emendamenti 3.1 e 3.2 andavano appunto nella direzione

L'approvazione di tali emendamenti sarebbe un bellissimo segnale di tutela nei confronti dei nostri giovani; un segnale importante soprattutto in questo momento storico in cui i bambini e gli adolescenti sono sempre collegati in Rete, dove possono trovare di tutto. Parliamo tanto di formazione e informazione e quegli emendamenti andavano proprio nel senso della formazione e dell'informazione corretta, della Rete in un modo corretto e non sbagliato. Il non accoglimento di tali emendamenti significa non volere veramente bene ai nostri giovani e ai nostri bambini; significa

si chiede di introdurre l'obbligo da parte dei *social network* di richiedere un documento d'identità all'atto dell'iscrizione dell'utente, ovviamente per poter a una più veloce identificazione del proprietario dell'*account* in caso di reati commessi sul *web.* Sappiamo che c'è anche una proposta a firma di Italia Viva che va in questa direzione, e quindi una proposta della maggioranza, depositata alla Camera, se non erro a prima firma dell'onorevole Marattin. Pertanto, non capisco perché non dare il via libera a un emendamento che mira a tutelare gli utenti del *web* da reati troppo spesso odiosi

Serve uno strumento di identificazione dei fruitori del *web*, che non può essere più una giungla dove tutto è permesso. Chiedo pertanto anch'io al Governo di rivedere la posizione su questo emendamento.

Grazie

Il rischio è che vengano pubblicizzati come cattivi i cibi del nostro *made in Italy*. Un esempio su tutti: un cibo ad alto contenuto di grasso come il parmigiano potrebbe essere indicato come cibo cattivo, con una pubblicità negativa. negativa. Su questo argomento l'Europa sta massacrando le nostre imprese, le nostre aziende, i nostri agricoltori, i nostri industriali. Noi stiamo

di latte e di trasformazione della carne. La scorsa settimana il non decidere del Parlamento europeo è stato gravissimo: un *hamburger* non è vegano, un *hamburger* è di carne. Sia chiaro. Non possiamo continuare a prendere in giro gli italiani, ma dobbiamo parlare in modo corretto e chiaro. La prima etichettatura - ricordatevelo - è la denominazione corretta di un prodotto, attraverso la sua identità, attraverso la sua catena produttiva e la sua filiera. Il ministro Bellanova tutti i giorni ci parla di aiuto alle filiere; vorremmo capire quali sono detti aiuti. Se l'Europa dà le risorse - come ha detto prima il Vice Ministro - sia chiaro che devono essere identificate bene, altrimenti si rischia di trovarsi di fronte a un parolaio collettivo da televisione, che non serve a nulla. Noi andremo in crisi; tutte le nostre imprese e il milione e mezzo di partite IVA agricole verranno a prendere a calci nel sedere chi di dovere. *(Applausi)*.

Signor Presidente, era molto tempo - non so quanto - che non esaminavamo un disegno di legge ordinario, con gli emendamenti e la dichiarazione di voto sull'articolo, che per fortuna non è stata ancora abolita da un decreto del Presidente

soprattutto in un momento di grande difficoltà per il mondo della cultura, dell'arte, dello spettacolo, della letteratura, al quale voglio inviare la piena solidarietà *(Applausi).* Il bavaglio alla cultura, al cinema e alla musica non risponde a esigenze di salute, stando ai dati statistici che sono stati divulgati, anche all'indomani del Festival del cinema di Venezia, della Festa del cinema di Roma e di eventi culturali importanti, che non hanno determinato un aggravamento della drammatica situazione in cui ci troviamo, anzi. Il maestro Muti in una lettera molto bella e importante, con l'equilibrio e l'autorevolezza del suo dire, al di sopra

varata. Contro questa direttiva europea c'è stato il peso delle *lobby* dei colossi della rete, adusi al saccheggio digitale: Google, Facebook, Amazon rubano i contenuti dell'arte e del sapere senza pagare la creatività. *(Applausi)*. Scrivere un romanzo, un'opera musicale o una canzone - anche la cultura popolare non va disprezzata - realizzare un film, produrre informazione televisiva, scrivere un articolo su un giornale

di operatori della cultura, dell'informazione, del giornalismo e della letteratura che non sono i grandi protagonisti che possono resistere anche un anno senza eventi, né concerti.

a Piazza del Duomo in maniera composta, portando quei bauli che in genere si usano quando si organizzano i concerti e le interpretazioni liriche. La tutela del diritto d'autore serve anche a quei lavoratori della cultura, della musica e dell'arte. Per questi motivi, siamo molto favorevoli

chiara. Se la cultura, l'arte e lo spettacolo vengono saccheggiati, noi uccidiamo la creatività, che deve essere remunerata e tutelata anche nell'epoca dell'elettronica avanzata e della digitalizzazione, che che devono essere un'opportunità per la conoscenza e non un furto del sapere legalizzato. È infatti questo che sta avvenendo. Onorevoli colleghi, su 4,5 miliardi di euro di volume di affari in Italia

conoscenza, ma anche riconoscimento della proprietà intellettuale e del diritto d'autore. L'articolo 3 del provvedimento - lo dico al Governo - non conclude l'*iter,* perché servono i provvedimenti attuativi.

solidarietà verso il mondo dell'arte, della cultura, della musica e dello spettacolo, di cui il Governo non si sta occupando affatto.

che va avanti da molto tempo. Chiede di porre una graduale esclusione dal 1° gennaio 2024 fino al dicembre 2030 degli obblighi di miscelazione

di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, come l'olio di palma. Ciò crea chiaramente un conflitto importante con l'uso agricolo dei terreni, che non solo è grave perché veniamo a perdere altro uso di terreno agricolo, ma anche perché, nel momento in cui c'è la trasmigrazione della produzione agricola, si vanno a produrre molte più

decisamente più corposo e la Commissione si è posta il problema di poter collocare - per esempio - gli impianti fotovoltaici anche sui terreni dell'*ex* discariche, su cui c'era una condivisione complessiva. Si è posta il problema di semplificare gli interventi sugli impianti anche quando vanno al di là della sostituzione delle batterie di alcune parti. Si è posta tutta una serie di passaggi.

attraverso il coinvolgimento dei consorzi. Non si capisce perché una parte della maggioranza abbia una preclusione ideologica rispetto al sistema consortile senza il quale il nostro Paese sarebbe molto più indietro in vari settori, compreso quello dei

"*Al comma 1 sostituire la lettera* dd) *con la seguente*: «prevedere la graduale esclusione, a partire dal 1° gennaio 2024, da completare entro il 31 dicembre 2030, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da materie prime o relativi residui e sottoprodotti derivati ad elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni»".

a valutare, nell'ambito della revisione della normativa di settore, una proroga del termine ultimo per l'entrata in esercizio

Colleghi, intanto vi dico che non è che improvvisamente abbiamo dei guasti. Avendo cambiato le modalità di intervento, alcuni microfoni

proprio l'evoluzione delle cosiddette energie rinnovabili. Chiediamo quindi che nel settore delle energie rinnovabili, anche in deroga a precedenti disposizioni normative, le cave, le discariche esaurite, le aree ripristinate dal punto di vista ambientale, a seguito di procedimenti di bonifica, ai sensi di quanto disposto dalla normativa, non siano considerate agricole, ai fini dell'ammissione agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a prescindere dalla qualificazione delle medesime, dettata dal pertinente strumento urbanistico. Questo per fare in modo che su terreni non più utilizzabili per nessun altro scopo possano invece insistere, con gli incentivi che meritano,

una richiesta di votazione per parti separate, chiedo all'Assemblea di pronunciarsi su questo punto.

l'emendamento 5.18 vuole riordinare la normativa vigente in materia di riconoscimento degli incentivi statali

realizzati su discariche chiuse, cave esaurite o siti di interesse nazionale o contaminati, che sono Queste tre tipologie di aree, alla fine della loro funzione, prendono la destinazione agricola. FER1 era in contrasto con il decreto-legge n. 1 del 2012, che di fatto vieta il riconoscimento degli incentivi per impianti fotovoltaici realizzati a terra su aree agricole. Questa discrepanza, che nel

il raggiungimento degli obiettivi per quanto riguarda le maggiori fonti di energia rinnovabili; non solo non avrebbe comportato un aumento

nell'ottica di una migliore transizione energetica, che non può che passare attraverso le città sostenibili. Ricordo a tutti i colleghi qui presenti che, durante gli oltre due mesi di *lockdown*, quando la mobilità si è praticamente ridotta a zero, tutti i fautori di quella elettrica si aspettavano un crollo delle emissioni di polveri sottili (PM10, PM2,5 o diossido di azoto). ambientale (ARPA) abbiamo registrato valori totalmente inalterati, a conferma che l'inquinamento atmosferico è prevalentemente prodotto dal riscaldamento domestico,

l'uso del teleriscaldamento efficiente, prodotto cioè con il calore di scarto dei processi industriali e con l'utilizzo di fonti rinnovabili. Non capiamo dunque i motivi di questa contrarietà: c'è un profondo pregiudizio, che si vede anche nel cosiddetto superbonus. Avete infatti introdotto il beneficio del superbonus per l'allaccio ai sistemi di teleriscaldamento efficiente solo nei Comuni montani oggetto di infrazione: è una presa in giro! *(Applausi)*. Dovremmo invece promuovere il tele riscaldamento efficiente in tutto il Paese

tantissime. I vantaggi del teleriscaldamento efficiente sono plurimi: certamente c'è una maggiore efficienza energetica, che è uno dei tre obiettivi

PM2,5, di ossidi di azoto; c'è più sicurezza nelle case, perché con il teleriscaldamento una famiglia toglie la caldaietta in casa, che ha necessità di manutenzione e controllo, a fronte di un impianto comune, e ci sono

Grazie

per lo sviluppo della capacità di generazione di energia da fonti rinnovabili che non sono comprese nel perimetro definito dal

La maggioranza è contenta perché in Europa il Consiglio europeo, la Commissione europea e il Parlamento europeo, quando si metteranno d'accordo, voteranno per un ulteriore taglio delle emissioni di CO2 nel 2030 (oggi è fissato a meno 40 per cento), perché si vuole raggiungere la neutralità climatica nel 2050.

sui tetti che avevano l'Eternit e sui nuovi impianti fotovoltaici o eolici, rispetto a un contingente di potenza incentivabile di 1.300 ne è stato richiesto in posizione utile meno di un terzo. Il problema di realizzare impianti da fonti di energia rinnovabile

le rinnovabili speciali (come geotermia, biogas, solare termodinamico e moto ondoso), il Governo non deve più dormire, perché c'è un'industria che vuole investire nella transizione energetica con i fatti e non con le parole e i numeri. Quindi non riusciamo a capire perché il Governo e la maggioranza vogliano votare contro questo emendamento, su cui la Lega invece voterà convintamente a favore.

chiediamo la verifica del numero legale. Il Senato è in numero legale.

Il senso dell'emendamento 5.310 è molto chiaro. Sapete tutti che la direttiva europea prevede che, per quanto riguarda gli obblighi di miscelazione di combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, ad oggi è ancora previsto l'utilizzo dell'olio di palma, che ha un impatto fortissimo (per quanto riguarda la deforestazione sappiamo quello che accade in Brasile e non solo). La direttiva prevede che dal 2024 ed entro il 2030 debba essere escluso dalla miscelazione l'olio di palma. Con Con questo emendamento prevedono un anticipo al 2023, come peraltro alcuni *player* nazionali stanno cominciando a fare.

il Governo considera l'ordine del giorno accoglibile con la seguente riformulazione nell'impegno: «a valutare l'opportunità, in sede di attuazione del regolamento UE 2018/1139 e di aggiornamento della disciplina nazionale in materia di volo da diporto e sportivo, di adottare ogni iniziativa che, compatibilmente con l'ordinamento eurounitario, favorisca lo sviluppo dell'industria del volo turistico italiana».

ancora che chi Io non lo sto verificando. Sono asimmetrici rispetto alle lucine, però è corretto. C'è poi il detto: «chi fa la spia non è figlio di Maria». Tre sono i presenti e tre sono i votanti. *(Commenti)*. Colleghi, collocatevi in modo che non ci siano questioni.

Colleghi, il distanziamento è una regola introdotta dai nostri senatori Questori, quindi se non vi collocate correttamente sospendo la seduta.

parere contrario su tutti gli emendamenti

Signor Presidente, sarò veramente succinto. Per me è molto interessante osservare come si stanno svolgendo queste dichiarazioni, considerando la materia degli articoli 10 e 11 della legge di delegazione europea, che riguardano argomenti piuttosto importanti. Le lugubri sigle che li contraddistinguono sono BRRD, CRD, CRR, SRM: sostanzialmente quello che va sotto il nome di pacchetto è quando vedo come stiamo analizzando qui in Aula queste disposizioni che capisco come è stato possibile che, per esempio, sempre in quest'Aula si siano approvate - peraltro, con una grande leggerezza da parte dell'attuale maggioranza - normative come quelle del *bail in*. Poi, naturalmente, è chiaro che esiste una saggezza della storia e su quel *bail in* il PD si è fatto del male e si sta facendo del male su altre cose. Per esempio, ho sotto gli occhi un meraviglioso titolo del dicembre 2018 in cui l'attuale ministro Gualtieri ci diceva che sui *non performing loan* in Europa era stato approvato un testo equilibrato. Quel testo equilibrato conteneva il famigerato *calendar provisioning*, che è quello che oggi, per esempio, il dottor Nagel, amministratore delegato di Mediobanca, definisce una bomba, e che fa preoccupare perfino il dottor Visco, governatore di Banca d'Italia, di cui all'epoca, però, non si rinvengono particolari opposizioni.

perché riguarda il tema del principio di proporzionalità che, senza entrare in dettagli tecnici inutili, si traduce in come non farci troppo del male nel recepire le normative europee. Quello che noi chiediamo è che non ci si avvalga della facoltà prevista dalla lettera *b)* del punto 145 dell'articolo 2 del regolamento 575/2013, in relazione in relazione alla soglia di 5 miliardi di euro del valore totale delle attività quale condizione ai fini della definizione di ente piccolo e non complesso. Richiediamo, cioè, che non venga abbassata la soglia al di sotto della quale una banca è considerata un ente piccolo e non complesso. Questo perché?

inevitabilmente incomberebbero su di loro se si decidesse di considerare piccola una banca con un capitale inferiore ai 5 miliardi di euro. Qui c'è fondamentalmente il tema del *gold plating*: gli altri Paesi non si avvarranno della possibilità di abbassare la soglia, quindi è assolutamente importante che anche noi chiediamo al legislatore delegato di non avvalersi della possibilità di abbassare la soglia, altrimenti, come al solito, andremo a competere in Europa con un braccio legato dietro la schiena. Per aver detto queste parole di saggezza, anche in altre circostanze, anche durante l'approvazione della BRRD nella prima versione,

Esattamente come accadde qualche anno fa al presidente Borghi di rivolgersi all'allora presidente del Consiglio Letta dicendo che non avevano capito cosa stessero facendo («Vi correranno dietro con i forconi e tiferò per gli inseguitori»), ed esattamente come ci siamo opposti, per esempio, al *calendar provisioning* così come magnificato da Gualtieri, qui chiediamo di fare attenzione. E se la storia ci ha dato ragione due volte, temo che ci darà ragione anche la terza volta. Auguri a questa maggioranza!

intanto dico di cosa si tratta. Qui si tratta, specificamente, di modificare la BRRD, ovvero la direttiva sulla risoluzione e i salvataggi salvataggi bancari, in Italia, si chiamano Etruria, Marche, Ferrara e Chieti, tanto per capire di cosa stiamo parlando e per ricordarlo affettuosamente ai nostri colleghi di maggioranza. dunque, lo specifico senso dell'intervento emendativo? Non mi diffondo: ci sono due punti e mi limito a ricordare il primo, in modo che

del potere di sospendere taluni obblighi e, in particolare, del potere di sospendere gli obblighi di pagamento. Chiediamo dunque che non venga esteso il potere di sospensione ai depositi ammissibili e in particolare che si introduca una clausola di salvaguardia, che assicuri un importo minimo giornaliero ai depositanti, al fine di mantenere la fiducia dei risparmiatori e la stabilità finanziaria, nelle circostanze eccezionali in cui si determini la necessità di attivare la sospensione dei pagamenti o il rimborso dei depositanti, cioè nel caso in cui si debba andare

ci sia un tema, che ritengo dovrebbe essere evidente a tutti. Forse non lo è, forse mi sbaglio e lo sottopongo

Il bagno di sangue fu un crollo del 60 per cento del comparto azionario in borsa, con tutto quello che sappiamo, in termini di danni ai risparmiatori e ai piccoli investitori. non era stata percepita la pericolosità dell'intervento legislativo che ci si accingeva a fare. Anni dopo, nel 2018, l'autorità bancaria europea (EBA) intervenne, dicendo che effettivamente la BRRD è un po' destabilizzante, dal punto di vista finanziario. In altre parole, l'Italia era stata usata come cavia, il *bail in* era stato applicato a casa nostra e a casa loro si disponevano risolutamente a non applicarlo. Del resto, gli sviluppi recenti in materia di *bad bank* europea ci suggeriscono che lì ci si accinge a salvare le banche con i soldi pubblici. A me non sembra che la lezione sia stata pienamente compresa, perché il semplice fatto che dobbiamo disporre un emendamento di questo tipo - che adesso la maggioranza boccerà - fa capire che la natura destabilizzante della normativa europea in materia di risoluzione di salvataggi bancari non è stata pienamente compresa dallo stesso legislatore europeo. Quindi ci aspettiamo altre copiose lacrime di coccodrillo dopo l'altro inevitabile incidente. Ci resterà la soddisfazione di averlo detto e voglio sperare che a lungo andare gli elettori si rendano conto che l'unica colpa degli economisti e, in generale, dei parlamentari della Lega non è non voler bene a mamma non voler bene a mamma Europa, ma è semplicemente capire un pochino prima quello che gli altri capiscono un pochino dopo. *(Applausi)*.

pubblica - mentre il Parlamento sta lavorando e il Senato è impegnato nella discussione e nella votazione di un disegno di legge di delegazione europea. Trovo tutto ciò inaccettabile e chiedo che il Senato sospenda immediatamente i lavori per consentire anche ai rappresentanti del popolo, quali noi siamo, di poter apprendere direttamente - se non di persona, almeno via Facebook o via televisione - quello che il presidente Conte riferisce agli altri ma non riferisce al Parlamento.

schermi il Presidente del Consiglio che fa l'ennesima conferenza stampa; probabilmente questa sera l'*audience* massima è a quest'ora, altrimenti l'avrebbe fatta più tardi. Riteniamo assolutamente indecente questo comportamento. Un comma, peraltro incostituzionale, approvato dalla maggioranza chiedeva di venire ad illustrare preventivamente *(Applausi)* i provvedimenti in Parlamento, non in televisione; davanti ai rappresentanti del popolo, non con Rocco Casalino.

nelle vite degli italiani *(Applausi)*, che sono stravolte da questi provvedimenti. Nelle piazze, purtroppo, c'è chi ha approfittato delle giuste proteste per infilarsi. Signor presidente Conte, se non viene da noi, saremo noi ad andare da lei.

Presidente, mi rivolgo anche ai colleghi della maggioranza per chiedere se non è frustrante essere in Aula mentre nelle piazze di mezza Italia, in quasi totale tranquillità... Ribadisco e ribadirò sempre che la violenza non è mai giustificata e non è mai la soluzione *(Applausi)*. Mentre noi siamo qui a votare...

al di là delle urla di qualche senatore nervoso del MoVimento 5 Stelle, che, mentre il Senato e la Camera stanno lavorando, il Presidente del Consiglio si faccia gli affari suoi in televisione. Non è accettabile, non è normale, è un insulto a milioni di famiglie e a milioni di lavoratori.

l'Italia col fiato sospeso, ci sono tassisti, commercianti, lavoratori della cultura e dello spettacolo, e noi siamo qui a votare. Alla Camera si sta votando sull'omotransfobia. Questo per darci l'idea di come qualcuno viva su Marte, mentre i problemi degli italiani sono i problemi di questa Terra Conte non è al Senato, non è alla Camera, ma in televisione. Senza Casalino, perché è a casa. Non è accettabile; andate avanti voi lavorare in questa maniera e a prendere in giro gli italiani. Noi usciamo da quest'Aula, perché il Senato ha ancora una dignità. Buon lavoro. E abbiate vergogna, se ne siete ancora capaci. Senatore Airola, lei ha i diritti e i doveri di tutti i senatori. Quindi si sieda e le verrà data la parola nell'ordine in cui l'ha richiesta.

Però - ahimè - il senatore Airola aveva decisamente ragione, perché sull'ordine dei lavori non ho capito che cosa ci abbia detto il senatore Salvini, oltre a parlare senza mascherina. mi permetta, signor Presidente: il suo richiamo mi è apparso un pochino tardivo. Ha lasciato volentieri che continuasse con un atteggiamento sprezzante delle regole del Senato. Dopodiché tutta questa messa in scena mi appare ridicola. Credo che sia corretto che ognuno di noi, soprattutto quelli che hanno incarichi istituzionali, faccia il proprio lavoro. Lo fa il Presidente del Consiglio e, tra i compiti del Presidente del Consiglio, c'è anche quello di informare tutto il Paese sui provvedimenti che il Governo sta prendendo. Il nostro dovere è fare le leggi e siamo qui a votare. Non credo che le due attività debbano necessariamente interferire. Però, guardi, parlo con grande spirito di collaborazione (è il messaggio che sto dando in queste ore al Paese, anche se mi sembra che le forze di centrodestra non siano affatto disponibili a riceverlo): se si chiede una sospensione, io sono favorevole alla sospensione. Senatore Marcucci, dopo aver dato la parola anche al senatore Airola, l'andamento dei nostri lavori e la richiesta di quattro interventi di fine seduta ci sta conducendo verso Grazie,

a portare avanti il nostro Paese soprattutto nei riguardi dell'Europa. *(Applausi)*. È vergognoso che si usi quest'Aula come il salotto di qualche *talk show* e lei non dovrebbe permetterlo. sempre equamente - e lo ricordo - lei ha fatto. Adesso noi dobbiamo finire di votare questo provvedimento e non ascoltare le

è un motivo per il quale certe cose devono comunque uscire) sia esattamente quello che non vuole in questo momento il popolo italiano. Non vuole che si strumentalizzi una seduta, non vuole che non si lavori, mentre questo è il risultato:

sta annunciando dei provvedimenti che il Paese attende e che non c'entra nulla con quello che sarà legittimamente il dibattito in quest'Aula. Ebbene, si è trovato un modo,

quando in realtà chi si dovrebbe vergognare è chi rinuncia a lavorare e a venire in Parlamento quando si tengono i lavori *(Applausi)*, è qualificante e direi in maniera potente riassuntivo del ruolo dell'opposizione del tutto accessorio rispetto alla

Guardate, vi state assumendo delle responsabilità gravi, perché non si può venire qui e fare gesti più o meno plateali, ad uso non so di chi, per poter fare un comunicato e soffiare sul fuoco, invece di assumersi tutti insieme delle responsabilità, ognuno certamente per la propria parte, noi come maggioranza e il

di un impoverimento del dibattito in Aula, perché gli spazi sono sempre più compressi. *(Commenti)*. Se non vi dà fastidio, colleghi, finisco, così la chiudo anche in fretta.

e questo comprimerà sempre di più gli spazi del dibattito parlamentare. Questa è una questione che pongo all'ordine del giorno un po' per tutti. Non volevo essere polemico con nessuno e credo di esserci riuscito.

previ accordi intercorsi, il calendario dei lavori della settimana corrente è integrato con i seguenti argomenti: informativa del Ministro dell'interno sui recenti disordini accaduti in alcune città italiane, domani alle ore 17; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, recante ulteriori misure per il contrasto della diffusione dell'epidemia da Covid-19, giovedì 29 alle ore 12,30

Giovanni, una persona mite e buona, ma soprattutto un professionista di grande valore. È stato portavoce alla Provincia di Roma e ha lavorato con Alitalia ed Equitalia.

Lazio. Una persona mite, competente, amata da tanti. Tutte le mattine mi faceva la rassegna stampa e avevo con lui un legame personale e profondo. Se n'è andato senza che la famiglia lo abbia potuto salutare. Oggi la bara è passata sotto la finestra di casa, da cui si sono affacciati la moglie e il figlioletto, che lo hanno salutato. portato al cimitero di Soriano nel Cimino, dove lo andremo a trovare nei prossimi giorni. Vorrei che anche in quest'Assemblea lui, che ha tanto collaborato, anche indirettamente, ai nostri lavori, fosse ricordato, così come lo è stato dalla stampa romana, laziale e anche nazionale, come un professionista buono, capace e competente. Ciao Giovanni, un amico vero. *(Applausi)*.

Signor Presidente, anche in Sardegna le terapie intensive, con l'aumento dei contagi da Coronavirus, sono già sature. Tuttavia, niente è stato fatto dalla Giunta sardo-leghista per far fronte al gravissimo problema della carenza cronica di medici e infermieri, il cui organico avrebbe dovuto avere un potenziamento. Il bando Il bando di qualche giorno fa per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna per personale medico da destinare a tutte le sedi ATS Sardegna per l'emergenza Covid-19 del 23 ottobre 2020, finalizzato alla formazione di un elenco di medici disponibili a svolgere attività assistenziale in Sardegna, oltre ad arrivare con un gravissimo ritardo, sebbene sia stato presentato dal Presidente della Regione come la soluzione a tutti i mali della sanità sarda, altro non è che un mezzo inadeguato, che difficilmente porterà nuove forze lavorative, men che anche meno provenienti da altre realtà regionali. Ciò a causa della scarsa attrattiva delle condizioni economiche proposte, decisamente inferiori a quelle offerte da altre Regioni italiane, penso ad esempio al Piemonte, che correttamente riconoscono degli incentivi allo svolgimento di prestazioni professionali gravose e rischiose come quelle dei reparti Covid-19. Non solo: le inerzie della Giunta sardo-leghista si sono veramente rivelate delle voragini, anche nel campo della scuola e dei trasporti. In Sardegna si è dato il via alle lezioni nella totale assenza di un programma che fosse in grado di conciliare il diritto allo studio con un adeguato sistema di trasporto pubblico a tutela della salute degli studenti e dei pendolari di tutta l'isola nell'emergenza coronavirus. Sono impresse nella nostra memoria l'immagine di tanti studenti sardi costretti a rimanere a terra, perché è rimasto invariato il numero degli autobus e quello delle corse, nonostante le regole anti Covid-19 impongano la riduzione delle presenze a bordo con limitato coefficiente di riempimento, e le scene dei mezzi sovraffollati dei ragazzi che indossano le mascherine, ma tra i quali è impossibile osservare il prescritto distanziamento. La giunta Solinas non è stata in grado di predisporre le misure necessarie a tutela della salute e del diritto allo studio, con un ritardo imperdonabile che ha sicuramente influito in modo significativo sulla diffusione dei contagi. Il Consiglio regionale ha approvato di recente una legge, la legge regionale n. 27 del 5 ottobre 2020, che stanzia dei fondi per implementare il numero di corse del servizio di trasporto pubblico degli studenti e dei pendolari e per il trasporto scuolabus, gestito dai Comuni. Si tratta, però, di una legge alla quale ancora non è stata data attuazione e che, nell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria, non è solo tardiva, ma rischia di essere inefficace. Insomma, una gestione, quella del governo di centrodestra sardo leghista, destinata a far pagare a caro prezzo l'emergenza sanitaria in Sardegna. *(Applausi)*.

con la partecipazione commossa di amici e colleghi del corso di laurea. Il rettore ha salutato con affetto la mamma e i familiari di Lorena e sottolineato che questo momento solenne, che poteva e doveva rappresentare il raggiungimento di un obiettivo, di un traguardo della vita professionale di Lorena, deve, comunque, dare un segno alla cittadinanza che il rispetto e il ricordo di una persona, di un essere umano deve superare la burocrazia e le pastoie che molto spesso ostacolano le azioni più semplici e partecipate della vita quotidiana. La sedia vuota nell'aula, che doveva essere occupata da Lorena per coronare il suo percorso di studi e il raggiungimento finale di un sogno suo e della sua famiglia, deve essere, per tutti noi, un momento di riflessione e di compartecipazione sentita al dolore immenso e alla tragedia immane che ha colpito la famiglia di Lorena, e possa, in parte, ricordare il suo entusiasmo e la sua voglia di apprendere e crescere professionalmente. Questa occasione è stato anche un momento per ribadire la necessità di combattere e contrastare, in tutti i modi e con tutti i mezzi a disposizione, condannando in maniera ferma e decisa, la grave problematica della violenza sulle donne, sia fisica che psichica, e l'assoluta necessità di norme e provvedimenti concreti, capaci di contrastarla. Va in questa direzione l'approvazione del cosiddetto codice rosso. Questa lotta, oltre che dal punto di vista giuridico e istituzionale, va attuata anche attraverso un percorso di maturazione culturale capace di coinvolgere la scuola, la famiglia, dando supporto e il dovuto risalto all'attività delle associazioni coinvolte attivamente e direttamente nella difesa e nel sostegno delle donne vittime di violenza, che spesso si realizza tra le mura domestiche, prima che le aggressioni ripetute e le loro conseguenze traumatiche sfocino nel dramma estremo dell'omicidio. dobbiamo dimenticare le tante vittime innocenti, la cui unica colpa è stata quella di innamorarsi della persona sbagliata. Rivolgo alla collega Lorena e alla sua famiglia questo ricordo.